ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, nonché del parere della Giunta per il Regolamento espresso nella seduta del 7 giugno 2006, all'attribuzione

ha riscontrato, nella seduta del 9 luglio 2009, che il candidato che segue immediatamente l'ultimo degli eletti nell'ordine progressivo della lista alla quale apparteneva il predetto senatore è Alberto Tedesco.

Onorevoli colleghi, con profondo dolore e grande commozione, comunico all'Assemblea odierna un nostro militare, il caporal maggiore paracadutista Alessandro Di Lisio, è morto e altri tre paracadutisti sono rimasti feriti quando una pattuglia della Folgore e del 1° Reggimento Bersaglieri è stata attaccata con un ordigno esplosivo, posizionato lungo la strada, a nord-est di Farah, in Afghanistan. È l'ennesimo tributo di sangue che il nostro Paese paga allo sforzo che la comunità internazionale sta compiendo per favorire il processo di pace in una regione difficile e martoriata da anni di guerra. Le nostre truppe sono in Afghanistan per una missione di pace e quindi per portare pace. Anche per onorare la memoria di chi ha dato la vita, è necessario proseguire questa missione internazionale in quelle difficili terre. Nei mesi scorsi ho potuto personalmente constatare la professionalità, l'impegno, la passione e lo spirito umanitario con cui i nostri soldati contribuiscono a questo delicato lavoro. Un lavoro che li vede impegnati in un'opera di ricostruzione di scuole, infrastrutture, centri sanitari per alleviare le condizioni difficili in cui vivono le popolazioni locali. Sono certo d'interpretare i sentimenti di tutti rivolgendo parole di commossa solidarietà e di profondo cordoglio ai familiari del militare caduto. Partecipiamo al grande dolore e ci stringiamo con affetto a tutti loro. Il nostro sincero cordoglio va naturalmente all'Esercito e alla Brigata Folgore. Ai tre paracadutisti rimasti feriti nell'attentato l'augurio di pronta e completa guarigione. Non posso non aggiungere il nostro rinnovato e sentito ringraziamento a tutti i militari che in Afghanistan, come in altre parti del mondo, continuano a portare avanti il loro difficile, quotidiano impegno per la pace e per la sicurezza dei popoli. In segno di lutto sospendo la seduta per 10 minuti.

Onorevoli colleghi, il 19 luglio 1992, in via D'Amelio a Palermo, la mafia, dopo 57 giorni dalla strage di Capaci, tornava a colpire il cuore dello Stato, uccidendo il giudice Paolo Borsellino e gli uomini di scorta della Polizia di Stato Agostino Catalano, Emanuela Loi, Eddie Walter Cosina, Claudio Traina, Vincenzo Li Muli. Un potente esplosivo, collocato all'interno di una FIAT 126 posteggiata dinanzi all'abitazione dell'anziana madre del giudice, seminava in pochi secondi morte e devastazione. Lo scenario agghiacciante di autovetture in fiamme, di palazzi circostanti la via profondamente danneggiati dagli effetti dell'esplosione non lasciava margini di dubbio sulla spietata volontà omicida degli attentatori. Oggi, a distanza di diciassette anni da quel tragico attentato, ricordiamo con grande commozione quei terribili momenti e onoriamo sei servitori dello Stato. Paolo Borsellino era entrato in magistratura a soli 23 anni, il più giovane giudice d'Italia. Dapprima pretore a Mazara del Vallo, poi a Monreale, nel 1975 era stato trasferito all'Ufficio istruzione di Palermo e, per volontà del consigliere istruttore Rocco Chinnici, era entrato a fare parte del *pool* antimafia, assieme, tra gli altri, a Giovanni Falcone. Se si possono sintetizzare con poche espressioni le qualità e le caratteristiche che si richiedono ad un magistrato, si deve parlare di profonda conoscenza delle leggi, di rigore, di vera autonomia, di capacità di conoscere la realtà dei fatti di cui ci si occupa e di saperli approfondire con assoluta obiettività, con grande competenza e profonda onestà. Paolo Borsellino rappresentava tutto questo; era pienamente consapevole della sua funzione di magistrato e della necessità di svolgerla avendo quale unico interesse il bene dello Stato. Dal momento in cui era stato trasferito a Palermo, aveva iniziato ad occuparsi di criminalità organizzata, accostandosi al tema con grande umiltà, ma anche con la ferma determinazione di riuscire a comprendere la struttura ed il modo di agire della mafia, nella piena convinzione che lo Stato e la magistratura dovessero porsi con determinazione dinanzi al fenomeno, dapprima per comprenderlo e quindi per contrastarlo. Per questo aveva iniziato a svolgere indagini sempre più incisive, in un'epoca in cui ancora non erano iniziate le collaborazioni con la giustizia, avvalendosi con grande scrupolo degli strumenti investigativi - ben diversi da quelli attuali - che il codice di allora consentiva. Proprio in quegli anni aveva visto cadere per mano mafiosa investigatori e magistrati a lui vicini: il vice questore Boris Giuliano, il capitano Basile, i commissari Montana e Cassarà, il consigliere istruttore Rocco Chinnici, il procuratore Gaetano Costa. Anni quelli di dolore, ma anche di grande volontà di andare avanti accantonando sensi di paura e di smarrimento, per riuscire a rendere libera la Sicilia. In costante simbiosi con Giovanni Falcone, Paolo Borsellino aveva concorso con la sua attività instancabile alla riuscita del primo maxiprocesso. "La gente fa il tifo per noi", aveva detto sentendo che quel processo che si stava organizzando per la prima volta veniva seguito e sentito dai siciliani come l'inizio di una nuova fase storica. Finalmente il popolo siciliano iniziava ad avere consapevolezza che la mafia, di fronte alla quale fino ad allora si era acquietato, non fosse più invincibile. Poi l'esperienza di Borsellino a Marsala come procuratore della Repubblica e, dal 1991, il ritorno a Palermo al posto di procuratore della Repubblica aggiunto, ricoperto fino alla sua morte. Borsellino era un magistrato di grande rigore, di grande serietà e professionalità, ma anche di grande umanità. Soleva dire che il giudice deve non solo apparire, ma soprattutto essere imparziale, senza mostrare mai all'esterno le proprie ideologie o i propri convincimenti politici. Così, spiegava, il magistrato si rende credibile ed autorevole. E si comportava di conseguenza. Uomo dai profondi valori religiosi, cattolico fervente e praticante, amava la sua famiglia oltre ogni cosa. Dedicava ai suoi figli tutti i momenti, seppur brevi, che riusciva a strappare al lavoro. E amava i giovani, la forza su cui contare per poter cambiare il futuro e le cose. Per questo non smetteva di andare nelle scuole a parlare dei veri valori, a raccontare agli studenti di mafia, dei mafiosi, dei metodi utilizzati per arricchirsi illegalmente, coinvolgendo i giovani con il suo dialogo chiaro e convincente, cercando di renderli partecipi e di fare loro comprendere i pericoli della droga. E cominciava ad accorgersi che stava per nascere nelle persone una nuova coscienza, che la gente comune, così coinvolta, aveva recepito questi sentimenti e intendeva divenire essa stessa protagonista della lotta alla mafia. Una vita, quella di Paolo Borsellino, interamente vissuta per lo Stato, per gli altri, per la sua terra, per un futuro migliore. Se oggi le cose cominciano a cambiare, se i risultati costanti nella lotta alla mafia si susseguono con ritmo incalzante, lo dobbiamo ad uomini come Borsellino, come Falcone, che hanno tracciato il percorso con il loro lavoro fino all'estremo sacrificio. Oggi commemoriamo un uomo al servizio dello Stato, della giustizia, delle Istituzioni. Ricordiamo gli agenti della Polizia di Stato, che per proteggerlo hanno sacrificato anche le loro giovani vite. Emanuela Loi è stata la prima donna della Polizia di Stato ad essere uccisa dalla mafia; assieme a lei gli altri quattro agenti, a cui va la nostra commossa riconoscenza. Il ricordo di Paolo Borsellino, eroe della legalità, e di tutti gli altri martiri caduti per mano mafiosa ha motivato ancor più l'attività antimafia del Parlamento, che non è mai stata così ferma e decisa. Ne sono prova tutti gli interventi legislativi emanati nel tempo e ancor di più quelli recentemente approvati, che hanno reso più efficace l'azione dello Stato contro ogni forma di criminalità organizzata. Anche le prossime leggi, in fase di discussione, intendono mantenere alta l'attenzione su questo fenomeno, con mezzi sempre più incisivi di contrasto. Lo Stato ha dimostrato di saper reagire e lo ha fatto con atti concreti; e lo continua a fare. E su questo tema tutti gli schieramenti hanno sempre collaborato costruttivamente, approvando normative sempre più efficaci all'azione di magistratura e forze dell'ordine. La lotta alla mafia è un patrimonio collettivo dell'intero Paese; è da sempre una priorità condivisa. Liberare il Sud dalla criminalità mafiosa significa dare respiro all'intero nostro Paese. Intervenire sull'esportazione illegale di capitali all'estero, impedire fenomeni di riciclaggio, aggredire i patrimoni mafiosi con misure di prevenzione sempre più mirate, colpire l'economia sommersa, braccio economico anche della criminalità organizzata, significa rafforzare il nostro mondo produttivo fondato sul vero e onesto lavoro e tutelare concretamente la legalità. Con questo fermo convincimento, potremo dire di aver onorato la memoria di Paolo Borsellino e di avere contribuito a creare un futuro migliore per le nuove generazioni.

la cui integrità non è mai stata scalfita, nonostante gli anni e le vicende trascorse. Un uomo la cui consapevolezza politica e culturale ha reso fondamentale quella difficile via del cambiamento per la lotta e il contrasto alla mafia. Nato e cresciuto a Palermo nello stesso quartiere di Giovanni Falcone - anche lui, lo sappiamo bene, ammazzato - e anche di Tommaso Buscetta, come in tanti quartieri non sarebbe stato difficile lasciarsi trasportare da cattive compagnie, piuttosto che crescere e studiare. Ma Paolo Borsellino no, Paolo Borsellino ha sempre avuto ben chiaro il concetto di legalità, ed è per questo che si è sempre battuto affinché questa venisse rispettata. La sua determinazione e la sua voglia di rendere migliore quella Palermo degli anni '60, afflitta dalle conseguenze di uno Stato invisibile ed assente, la sua tenacia nella ricerca della verità, fino ai limiti dell'ostinazione, sono sempre state le sue prerogative. Voleva mettere a disposizione di quella terra, tanto amata e odiata al contempo, la sua forza intellettuale e professionale per renderla migliore. «La lotta alla mafia, primo problema morale da risolvere della nostra terra bellissima e disgraziata» - diceva «non deve essere soltanto una distaccata opera di repressione bensì un movimento culturale e morale». Significava smuovere le coscienze, rompendo quel sentimento di accettazione della convivenza con la mafia che ne costituisce la sua stessa forza. Paolo Borsellino, e insieme a lui tanti altri, ci ha creduto veramente. È sempre stato uno che conosceva e riconosceva nei diritti delle persone la giusta via verso la legalità, la giusta via verso la democrazia e la giustizia. Tutti conosciamo la sua storia, la sua vita (un vero e proprio atto d'amore verso la sua terra), le sue imprese giudiziarie, le inchieste condotte insieme all'amico fraterno e collega, il giudice Giovanni Falcone (la cui morte non arrestò il suo impegno civile, anzi, lo spinse a lavorare di più), le inchieste che condussero insieme, che portarono ad un vero e proprio smantellamento della criminalità organizzata, siciliana e non. Tutti sappiamo bene con quanto impegno e con quanto amore svolgesse il suo lavoro, pur rinunciando alla sua famiglia e ai suoi affetti più cari, cosa di cui si rimproverò fino alla fine dei suoi giorni: «Se non fosse per il dolore di lasciare la mia famiglia potrei anche morire sereno», disse una volta partecipando ad un incontro organizzato pochi giorni prima della sua morte. quell'incontro parlò della sua condizione con la fredda consapevolezza di un condannato a morte: sapeva benissimo di essere un «morto che cammina», di essere nel mirino di Cosa nostra e che difficilmente la mafia si sarebbe lasciata scappare quella vittima ormai designata da tempo. Questo oggi potrebbe essere il motivo per cui qualcuno potrebbe erroneamente pensare che la sua vita non sia servita a molto, visto che la mafia è ancora uno dei «cancri» della nostra società.

In quella calda giornata siciliana la mafia ha creduto di avere ucciso, e dunque eliminato, l'ennesimo "bastian contrario" di una Palermo che stava diventando sempre più ingombrante ed importante anche a livello nazionale. Quel giorno oltre a perdere una persona straordinaria, un magistrato attento e capace, un uomo sensibile che ha speso tutta la sua vita senza mai esimersi o scoraggiarsi davanti ad alcuna difficoltà, i suoi figli sono stati privati di un padre. Ma, sopra ogni cosa, abbiamo perso l'uomo che insieme a Giovanni Falcone, insieme a Peppino Impastato, insieme a Boris Giuliano, a Carlo Alberto Dalla Chiesa, a Ninni Cassarà, a Libero Grassi, a Claudio Domino (un bambino di soli 11 anni, la cui unica colpa è stata quella di aver assistito ad un sequestro di persona),

all'infinito: l'elenco delle vittime della mafia è lunghissimo e parla di innocenti, di persone comuni, di imprenditori, di bambini, di intere famiglie annientate e distrutte dal dolore, perché in tutte quelle stragi sono stati segnati per sempre i destini e le vicende di quelle famiglie. Di persone come Borsellino non possiamo che essere profondamente orgogliosi. Sono patrimonio del nostro Paese. Le loro vite, i loro sacrifici non solo sono stati l'inizio di una perseveranza nella speranza di un mondo migliore, ma sono stati anche la ricerca e la voglia di giustizia. Oggi, oltre al giudice Borsellino però, il nostro ricordo deve andare anche agli uomini della sua scorta coinvolti nella strage di via D'Amelio e a tutte le persone e le famiglie vittime di mafia. Perché quel ricordo viva per sempre. *(IdV)*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, signori rappresentanti del Governo, è sempre una forte e dolorosa emozione per un palermitano ricordare ciò che accadde quel giorno di 17 anni fa: in molti in città sentimmo il terribile boato dell'esplosione alle ore 16,55 del 19 luglio e in molti, io tra questi, pur non sapendo ancora cosa fosse successo, ripensammo alla strage di Capaci di poche settimane prima, quando le strade di Palermo si riempirono di auto della polizia, autoambulanze, Vigili del fuoco, e nell'aria non si sentiva altro che il sinistro urlo delle sirene. Purtroppo, quell'inquietante sensazione che la mafia avesse di nuovo colpito si rivelò drammaticamente esatta. Pensate, due uomini quasi coetanei, separati solo da un anno, nati nello stesso quartiere della Palermo araba, la Kalsa, in due case separate solo da un centinaio di metri, accomunati dalla voglia di lottare per una Sicilia finalmente libera dal giogo mafioso e per uno Stato realmente democratico, libero a sua volta da ogni tentazione di connivenza ed impermeabile ad ogni tentativo di infiltrazione. Già nel 1985 la mafia aveva emesso la sentenza di morte nei confronti dei due magistrati, l'anno in cui vennero uccisi i commissari Giuseppe Montana e Ninni Cassarà, i loro stretti collaboratori. Dopo pochi minuti la notizia che si era compiuta un'altra strage di mafia, in cui era rimasto ucciso il giudice Paolo Borsellino, si diffuse in tutta Palermo, la Palermo del cardinale Salvatore Pappalardo. Ricordate ai funerali del generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, ucciso insieme alla moglie Emanuela Setti Carraro e all'agente Domenico Russo, il 3 settembre 1982, la frase pronunciata dal cardinale Salvatore Pappalardo: «Povera la nostra Palermo!». Forse da lì, da quella frase del proprio pastore, cominciò il cammino di riscatto dei palermitani e dei siciliani (che poi culminò anni dopo con le catene umane e le lenzuola ai balconi per dire no alla mafia), che solo un giorno prima, sul luogo dell'eccidio, avevano lasciato un cartello con scritto: «Qui è morta la speranza dei palermitani onesti». Cosa era cambiato dopo quel grido di dolore lanciato ben dieci anni prima, nel 1982? Ancora sangue: il 23 maggio del 1992 Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo e gli uomini della scorta Vito Schifani, Rocco Di Cillo, Antonio Montinaro; poco dopo, il 19 luglio, il giudice Paolo Borsellino e gli addetti alla scorta Agostino Catalano, Emanuela Loi, Vincenzo Li Muli, Eddie Walter Cosina e Claudio Traina; un anno dopo, la barbara uccisione di padre Pino Puglisi. La strana sensazione che si fosse sotto una cappa di terrore che copriva l'intera città l'avemmo qualche settimana prima, nell'ultima apparizione pubblica di Paolo Borsellino. Il 25 giugno, durante un incontro organizzato alla Biblioteca comunale di Palermo, Paolo Borsellino era già cambiato: il suo tono era basso, i lineamenti del suo volto tirati e lui, sempre padrone dei suoi sentimenti (come si può notare nelle varie interviste concesse),

Io c'ero nell'atrio di quella biblioteca e non dimenticherò mai la strana sensazione, che abbiamo avuto in tantissimi, che il prossimo bersaglio non poteva essere che lui, sperando che lo Stato riuscisse a proteggerlo. La strage di via d'Amelio, dopo quella di Capaci, sembrò un'ulteriore affermazione dello strapotere assoluto della mafia, ma anche il segnale che qualcosa s'era rotto, pure all'interno dell'organizzazione criminale, dopo la presa del potere da parte dei corleonesi nella lunga e silente strategia del sotto traccia, dell'infiltrazione nei gangli dello Stato e delle istituzioni. Una strage, quella che ha ucciso Borsellino, avvolta in troppi misteri. Una strage, come accaduto per tanti altri misteri nella storia della nostra Repubblica, su cui non è ancora stata raggiunta una verità vera. Sarebbe troppo lungo elencare fatti ed episodi che, ormai, sono agli atti dell'inchiesta giudiziaria ancora in corso. Qualcuno forse sta pensando che in una commemorazione bisogna parlare solo delle alte qualità qualità del commemorato, ma noi pensiamo diversamente. Farei un grande torto ad un uomo come Paolo Borsellino, uomo-eroe, se non parlassi del contesto criminoso di quegli anni, soprattutto di ciò che lo ha ucciso e dei valori in cui credeva e per cui, consapevole, ha dato la vita. Consapevole, sì. Ricordate la sua terribile frase dopo la morte dell'amico e collega Falcone: «Io sono un morto che cammina». Non poteva essere più consapevole di così, eppure non è fuggito, ha continuato a lottare contro un'organizzazione criminale, ma anche, come da sempre, contro le collusioni tra mafia e politica, tra mafia e finanza, tra mafia ed economia, tra mafia e pubblica amministrazione. Lo ha fatto almeno fino a quel tragico pomeriggio, quando stava compiendo un atto umanissimo: stava andando a rendere visita a sua madre, alla sua famiglia. Distratto lo Stato che non aveva pensato, dopo Capaci, di mettere in sicurezza quella strada frequentata dal giudice. C'è solo un modo, onorevoli colleghi, per ricordare Paolo Borsellino e Giovanni Falcone, nomi che non riesco mai a disgiungere, insieme a quelli di tutti coloro - giudici, uomini e donne delle forze dell'ordine, giornalisti, imprenditori, sacerdoti, gente comune - che hanno perso la vita per mano mafiosa: essere accanto alla magistratura che, insieme agli organi inquirenti, tanta strada ha fatto (anche se ancora tanta ne resta da fare) fare) per debellare questo cancro della nostra società; porre tutto il sistema della giustizia nelle migliori condizioni per lavorare, con uomini e mezzi sufficienti; fare leggi che aiutino le indagini e non quelle che le rendono più difficili; aiutare concretamente tutti coloro che, nell'ambito del proprio lavoro e della propria attività, dicono no al *racket*, al pizzo, alla sopraffazione; ma soprattutto - non meravigliamoci - coniugare nuovamente i binomi etica e politica, etica ed economia. Così vogliamo ricordare Paolo Borsellino, Emanuela Loi, Agostino Catalano, Vincenzo Li Muli, Walter Cosina e Claudio Traina. *(Applausi Signor Presidente, colleghe e colleghi, sono trascorsi 17 anni dalla morte, quel 19 luglio del 1992, del giudice Paolo Borsellino, ma stranamente sembra che non sia passato tutto questo tempo,

Nel 1963 Borsellino vince il concorso in magistratura, e credo sia necessario un grande amore per la propria terra, per la giustizia, per fare il magistrato in una terra difficile come la Sicilia. Nel 1975 Borsellino viene trasferito presso il tribunale di Palermo e a luglio entra nell'Ufficio istruzione processi penali sotto la guida di Rocco Chinnici. Nel 1980 arriva l'arresto dei primi sei mafiosi. Nello stesso anno il capitano Basile, suo collaboratore, viene ucciso in un agguato. Per la famiglia Borsellino, con l'arrivo della prima scorta, cambia la vita, con le difficoltà che ne conseguono.

Gli anni Ottanta sono gli anni del *pool* antimafia, che comprende tra gli altri Falcone e Borsellino, che lavorano sotto la guida di Rocco Chinnici, in seguito trucidato anche lui dalla mafia. Nel 1987 il giudice Caponnetto, succeduto a Chinnici, è costretto a lasciare la guida del *pool* antimafia per motivi di salute. Tutti a Palermo aspettano la nomina di Falcone al suo posto, e anche Borsellino è ottimista. Presto, però, si rende conto che il Consiglio superiore della magistratura non è dello stesso parere e in Borsellino prende corpo il terrore di veder distruggere il *pool*.

convoca Borsellino, che rinnova accuse e perplessità. È tutto inutile, perché il Consiglio superiore della magistratura non assegna il posto a Falcone. Cominciano a parlare i pentiti e le indagini su connessioni tra mafia e politica iniziano a prendere forma. Borsellino è convinto che per sconfiggere la mafia i pentiti abbiano un ruolo fondamentale. Anche i giudici però dovranno essere attenti. Controllare e ricontrollare ogni dichiarazione, ricercare riscontri ed intervenire solo quando ogni fatto può essere provato. Da questo momento in avanti gli attacchi a Borsellino, vista la sua posizione nei confronti del tribunale palermitano, sono incessanti. Comincia il dibattito sull'istituzione della superprocura e su chi porre a capo del nuovo organismo. Chiaramente, Borsellino vede in Falcone la persona ideale, ma nel maggio 1992

in questo momento che la mafia lo colpisce in via D'Amelio e lo uccide. Non c'è dubbio che gli attentati a Falcone e a Borsellino abbiano segnato in Italia un punto di svolta nell'atteggiamento della popolazione verso la mafia. Da allora, centinaia di migliaia di persone

Il senso dell'esistenza di Paolo Borsellino, come di molti altri che hanno pagato con la vita le loro scelte, è proprio questo: non vi è nulla di invincibile, tanto meno la mafia, con tutto quello che questo sostantivo significa. infatti, significa schiavitù, ingiustizia, arretratezza culturale e civile cui, per dirlo con le parole di Borsellino, si può sempre opporre il fresco profumo della libertà, che fa rifiutare il puzzo del compromesso morale, dell'indifferenza, della contiguità e, quindi, della complicità. Personalmente, mi rimane un unico rimpianto: non averlo conosciuto.

sono morti nella strage di Capaci e poi nella strage di via D'Amelio, ricordando le parole di chi è stato il maestro di tutti noi, Antonino Caponnetto. Recandosi a Palermo dopo la morte di Paolo Borsellino, Caponnetto disse: «Queste sono le parole di un vecchio ex magistrato che che è venuto, nello spazio di due mesi, due volte a Palermo con il cuore a pezzi a portare l'ultimo saluto ai suoi figli, fratelli, amici, con i quali ho diviso anni di lavoro, di sacrificio, di gioia ma anche di amarezza. Il ricordo è per l'amico Paolo, per la sua generosità, per la sua umanità, per il coraggio con cui ha affrontato la vita e con cui è andato incontro alla morte annunciata, per la sua radicata fede cattolica, per il suo amore immenso portato alla famiglia e agli amici tutti. Era un dono naturale, che Paolo aveva, di spargere intorno a sé amore. Ricordo ancora il suo appassionato e incessante lavoro, divenuto frenetico negli ultimi tempi, quasi che egli sentisse incombere la fine». Nel corso di questa preghiera, laica, ma fervente (come la definì), Caponnetto si rivolgeva al Presidente della Repubblica e gli diceva: «La gente di Palermo e dell'intera Sicilia, Presidente, ti ama, ti rispetta e, soprattutto, ha fiducia nella tua saggezza e nella tua fermezza. Paolo è morto servendo lo Stato in cui credeva, così come prima di lui Giovanni e Francesca. Ma ora questo Stato, che essi hanno servito fino al sacrificio, deve dimostrare di essere veramente presente in tutte le sue articolazioni, sia con la sua forza che con i suoi servizi. giunto il tempo, mi sembra, delle grandi decisioni e delle scelte di fondo. Non è più l'ora delle collusioni, degli attendismi, dei compromessi e delle furberie. Dovranno essere, Presidente, uomini credibili, onesti, dai politici ai magistrati, a gestire, con le tue illuminate direttive, questa fase necessaria di rinascita morale». Io credo che questo testamento, che ci ha lasciato Antonino Caponnetto, sia quello che quest'anno ha ripreso il presidente della Repubblica Napolitano recandosi a Palermo. Parlando della morte di Borsellino e di Falcone, il presidente Napolitano ha messo in luce che la mafia e le altre organizzazioni criminali hanno subìto profonde evoluzioni e trasformazioni, assumendo nuove fonti delittuose di arricchimento e di estensione del loro potere. Lo Stato democratico, come ha messo in luce il Presidente, deve quindi procedere decisamente oltre i rilevanti successi conseguiti anche di recente; deve fronteggiare la mafia e le altre organizzazioni criminali in tutte le espressioni: quelle tradizionali tuttora operanti e quelle nuove inserite in un contesto mondiale del tutto mutato. Sappiamo che contano altri importanti elementi per sconfiggere la mafia e la criminalità in Sicilia e nel Mezzogiorno. Contano la qualità della politica, il prestigio delle istituzioni democratiche, l'efficienza e la trasparenza delle pubbliche amministrazioni. Conta la crescita della coscienza civica e la fiducia nello Stato di diritto. Ed ecco il 19 luglio 1992. Un'autobomba mafiosa uccide, in via d'Amelio, Paolo Borsellino e gli agenti della scorta. Da servitore dello Stato Paolo Borsellino ha vissuto gli ultimi giorni della sua vita con la consapevolezza che la sua fine era prossima dopo, appunto, un'altra strage, quella di Capaci del 23 maggio 1992. Ho avuto l'onore di conoscere sia Giovanni Falcone che Paolo Borsellino. Il giorno della strage di Capaci ero al telefono con Paolo Borsellino, che si trovava sul luogo della strage. Paolo mi disse: «Spero che Francesca si salvi», e io gli dissi: «Mi auguro che Francesca non si salvi». Non avrebbe potuto sopravvivere alla morte di Giovanni. Successivamente, due giorni prima che Paolo Borsellino morisse, ero al telefono con lui e con Piero Vigna. Parlavamo della possibilità di interrogare insieme Gaspare Mutolo. Quest'ultimo si era pentito nelle mani dei magistrati di Firenze e voleva parlare soltanto con Paolo Borsellino. Fu un momento molto difficile. Paolo mi disse: «Forse vado in Germania perché devo chiudere una pista mafiosa; se non vado in Germania, sicuramente lunedì vengo a sentire Mutolo insieme a voi». Purtroppo la domenica Paolo Borsellino morì. Chi era Paolo Borsellino? La definizione più calzante: un eroe borghese, proprio come Giorgio Ambrosoli, un uomo, un magistrato che lascia un insegnamento di passione civile praticata nel luogo di lavoro dove la scelta o un caso ti portano ad operare e dove devi fare fino in fondo la tua parte, pur sapendo che può portarti alla morte. Come si comporterebbe oggi? Con il solito senso dello Stato, ma con fermezza, continuando a lavorare anche nelle condizioni più difficili, pronto a denunziare, anche pubblicamente, l'insufficienza delle istituzioni e a difendere la legalità e i valori della Costituzione. Non è necessario provare ad indovinare il suo pensiero. Sulla giustizia e sul pentitismo i suoi interventi sono lucidi e attuali. Basta leggerli. Il calo di tensione nella lotta contro la mafia, il nodo mafia-politica,

Un'organizzazione che si adegua costantemente ai tempi, anzi spesso la precede. La mafia in Italia sarà sconfitta solo quando avremo un'etica pubblica come quella di altri Paesi civili dove un politico, se coinvolto in affari criminali illeciti, scompare per la vergogna e per la impossibilità di sostenere la riprovazione sociale. Ho apprezzato, signor Presidente, le sue parole. Questo desiderio di voler combattere congiuntamente la mafia la onora ed io penso che lei onorerà questo impegno. Ci sono leggi molto serie in discussione. Queste leggi, se approvate, indebolirebbero moltissimo la lotta contro la mafia ed io sono convinta che potremo fare fronte comune contro questo. Non potremmo onorare la memoria di Borsellino e di Falcone se facessimo approvare leggi che indeboliscono la lotta contro la mafia, che non adeguano ad una criminalità

come fece quando Falcone non fu nominato alla Procura nazionale antimafia, come fece tutte le volte che voleva denunziare qualcosa che nelle pubbliche istituzioni non andava, e come fece andando alla morte nella consapevolezza, forse, che anche lo Stato poteva averlo abbandonato. Vorrei rivolgere un pensiero affettuosissimo: Borsellino e la sua famiglia erano miei amici. A Lucia, a Manfredi, a Fiammetta, a Agnese e a Rita Borsellino che combatte da anni una battaglia contro la mafia che onora la famiglia Borsellino, come Manfredi, tutt'oggi funzionario dello Stato, poliziotto, che continua l'attività di suo padre. Penso che a Borsellino dobbiamo rivolgere un grande ringraziamento, come a Giovanni Falcone. Lo dobbiamo però dimostrare nei fatti e dobbiamo pretendere che quella verità giudiziaria, cui faceva cenno anche il collega Giambrone, possa essere veramente raggiunta.

Signor Presidente, la ringrazio per aver voluto dedicare l'apertura della seduta odierna al ricordo di Paolo Borsellino e, come giustamente ha fatto, della sua scorta. Infatti, queste tragiche vicende, che hanno scandito in modo orribile e indelebile la storia italiana degli anni '90, hanno visto vittime non solo negli eroici magistrati - ed è inevitabile accostare il ricordo di Giovanni Falcone e di tanti altri rappresentanti dello Stato a quello di Paolo Borsellino - ma anche in tanti carabinieri, poliziotti, uomini e donne, nel tentativo - ahimè vano - di difendere la vita di chi tanto ha prestato la sua opera per la sicurezza di tutti noi. Credo quindi sia necessario che le istituzioni

- che nei giorni scorsi in Parlamento, nell'Aula del Senato c'è stato il voto finale, sono diventate leggi dello Stato nuove ed ulteriori norme antimafia,

dedicato una parte importante al sequestro e alla confisca dei patrimoni mafiosi, attività in corso da tempo ma che necessita sempre di strumenti più immediati, più penetranti; una scelta politica che

Credo pertanto che il Parlamento faccia bene, in queste occasioni, a dedicare parole di ricordo e di impegno politico e istituzionale, affinché non siano solo retoriche le parole che ricordano il sacrificio di chi non c'è più.

cogliere aspetti polemici. Sono convinto non solo che i fatti parlino per le leggi fatte, ma anche per quelle che si faranno, tutte improntate al rigore, alla necessità di concentrare l'iniziativa giudiziaria contro tutti i fenomeni di illegalità, ma soprattutto contro contro quei fenomeni mafiosi che tanto hanno avvelenato ed avvelenano la vita della Repubblica. Sono intervenuto anche perché ho un ricordo personale di Paolo Borsellino. responsabile dell'organizzazione giovanile del mio partito e, attraverso la disponibilità dell'onorevole Pippo Tricoli e di altri esponenti del mio partito, che da sempre condividevano un'amicizia

Mi colpì il fatto che la sera prima, il 29 settembre, arrivò a Siracusa alla guida di una macchina senza particolari misure di difesa. Lo accolsi e gliene chiesi la

Successivamente gli eventi e la strage di Capaci imposero misure di maggiore tutela che - ahimè, come lei stesso ha ricordato - non impedirono quanto avvenne: lo scempio, la potenza tragica, orribile e militare di quell'attentato mafioso, di un atto bellico che tutti ricordiamo in quelle immagini di strade e palazzi devastati. Ci colpì quell'esempio di grande rigore e semplicità: il fatto

e disse a quella platea di giovani militanti di destra - sapeva benissimo dove si trovava - che occorreva grande rigore. Molti di noi erano già consiglieri comunali o giovani esponenti nelle amministrazioni locali. mantenere grande rigore e pronunciò una frase che mi è rimasta impressa per tutta la vita: ragazzi, non rinunciate ai vostri ideali e portateveli dietro fino a quando non avrete i capelli bianchi. Gli anni sono passati, molti capelli bianchi sono spuntati, ma credo che il rigore nella lotta ai fenomeni criminali resti forte, anche sulla base di un insegnamento che molti di noi vivono come esperienza quotidiana, come scelta di campo per la legalità e la lotta alle mafie, con grande e profonda convinzione, anche per gli esempi che ci toccò di vivere da vicino e la semplicità con cui si affrontavano già nel 1990 fenomeni enormi. Voglio concludere ricordando una delle tante le frasi che sono state citate in questi anni e che Paolo Borsellino una volta ebbe modo di pronunciare: a fine mese, Grazie, di tutti gli italiani. Ricordare il suo esempio credo che sia non soltanto un dovere per noi, ma il modo per additare a tutte le generazioni un autentico eroe civile del nostro tempo, un esempio a cui guardare in ogni momento e in ogni istante della nostra opera di legislatori.

Esponente di spicco del Partito Repubblicano Italiano, nel 1975 ne divenne segretario nazionale. Con Oddo Biasini scompare l'ultima grande figura del repubblicanesimo storico, in cui aveva portato le caratteristiche tipiche dei repubblicani di tradizione romagnola, quella da cui provennero alcuni grandi esponenti repubblicani fra la fine dell'800 e il secondo dopoguerra, come Giuseppe Gaudenzi, che fu fra i fondatori del PRI nel 1895, Ubaldo Comandini e Cino Macrelli. Da loro proviene una grande tradizione amministrativa improntata a una fortissima passione politica, un assoluto disinteresse personale, il senso del dovere verso le istituzioni, un amore di stampo risorgimentale per l'Italia, un legame indissolubile per il proprio partito. Per gli uomini che vengono da questa tradizione, la politica è, prima di tutto, come aveva insegnato Mazzini, un apostolato popolare, un apostolato che Oddo Biasini ha esercitato nel corso intero della Recentemente, la Fondazione Ugo La Malfa ha pubblicato parte dei suoi diari, e di queste pagine vorrei portare alla vostra attenzione quella scritta il giorno della morte di Ugo La Malfa in cui Oddo Biasini, nonostante la lunga esperienza politica e a dispetto di chi dice che la politica indurisce i cuori, rivela i tormenti che attanagliavano il suo animo e manifesta quella consapevolezza del limite che solo le persone autenticamente e intellettualmente oneste hanno.

Grazie, che non desideravo, che temevo: Segretario nel 1975; riconfermato nel 1978: trascinato sempre riluttante ad impegni più forti delle mie capacità e soprattutto estranei ormai ai miei desideri. Ed ora la scomparsa di La Malfa dà una drammatica svolta alla mia vita politica. Mi manca la lena, ma sento imperioso il richiamo del dovere e non mi sottrarrò certo ad esso: ma quali saranno gli sbocchi di questa terribile responsabilità? A volte temo di essere travolto» «Come si concluderà questa vicenda? Mi domando a volte quali tempi mi stiano a fronte, e mi smarrisco». La sofferenza e il tormento che emergono dalle parole di Oddo Biasini sono la prova evidente di quanto egli, pur avendo raggiunto nel corso della sua carriera politica i traguardi più alti, avesse mantenuto una commovente semplicità d'animo unita ad un profondo senso di responsabilità e di rispetto per le Istituzioni che era stato chiamato a servire.

forti memorie personali e familiari al bellissimo ricordo di Oddo Biasini che è stato tracciato dalla senatrice Bianconi, non certo per completarlo, perché credo che quella bellissima citazione del suo diario, scritta il giorno della morte di Ugo La Malfa, sia il modo più degno per ricordarlo in questa Assemblea,

alla moglie e al figlio che rimane, ricordo quanto quest'uomo fosse stato provato, a 92 anni e già sofferente, quando, poco prima di Natale, gli era capitata

Dopo l'illustrazione, ciascun Gruppo avrà a disposizione 20 minuti, comprensivi degli interventi in discussione e in dichiarazione di voto. Ha facoltà di parlare il senatore Camber per illustrare tale mozione.

Per ultima, ci aveva sollecitato ad un'iniziativa sul tema delle condizioni della liberazione di Gilad Shalit la comunità italiana a Gerusalemme, che avevamo incontrato nel corso della missione che la Commissione per i diritti umani aveva svolto a Gaza, in Cisgiordania e in Israele. Come i colleghi sanno, Gilad Shalit è stato rapito più di tre anni fa. È stato preso non mentre partecipava ad uno scontro, non durante un'azione di combattimento, non durante un'azione repressiva, ma mentre svolgeva un presidio dentro i confini israeliani, in un'azione ordinaria Il suo rapimento è stato un'azione premeditata a freddo, e da allora nessuno lo ha visto. I familiari non ne hanno notizie nessuno ha potuto accertare il suo stato di salute. Si dice, ma anche questo non è sicuro, che forse suo padre sia riuscito a fargli arrivare un paio di occhiali, visto che i suoi erano stati rotti durante l'azione del rapimento. Tutte le norme sancite dal diritto internazionale, le norme che salvaguardano anche nel mezzo delle guerre l'inviolabilità del nucleo umano di ogni persona, sono state ignorate: nessuna delle garanzie che proteggono la vita e la dignità di un prigioniero è stata rispettata. Credo che su questo punto la comunità internazionale e anche una grande istituzione come la Croce Rossa abbiano fatto troppo poco e portino qualche responsabilità. Certo, la vicenda di Gilad Shalit s'intreccia con la storia degli ultimi tre anni, la storia della guerra in Libano fino all'operazione «Piombo fuso» a Gaza. È una storia terribile. Siamo stati a Gaza e abbiamo osservato la quantità e l'ampiezza della distruzione; siamo stati a Sderot e abbiamo visto le conseguenze dei missili, non solo sui morti che hanno provocato, ma anche sul clima che hanno costruito; siamo stati a Hebron e abbiamo sentito, abbiamo sentito, e seguito, che sono in corso negoziati. Abbiamo saputo di queste trattative, che tante volte sembravano vicine a un risultato e poi sfumavano; abbiamo sentito parlare di un possibile scambio di prigionieri e, di volta in volta, visto questa possibilità vanificarsi. Siamo uomini politici sappiamo che forse la sorte di Gilad Shalit è anche legata a quella del negoziato per la pace. Tuttavia, anche se sappiamo tutto questo c'è qualcosa in noi che si ribella all'idea che un giovane uomo, un ragazzo possa essere trattato come un oggetto, che l'unico suo valore risieda in quello che può essere scambiato con lui, come se la sua umanità fosse un dettaglio irrilevante. Per questo, mentre sosteniamo l'urgenza di una soluzione politica che apra la strada alla costruzione della pace, mentre riaffermiamo le nostre convinzioni su una soluzione che debba essere ricercata su quella linea che ormai la comunità internazionale ha consolidato e che riassumiamo nell'assunto «due popoli, due Stati», mentre riaffermiamo la necessità di un più forte impegno

ed ancora prima di consentire che siano garantiti a lui e alla sua famiglia quei diritti elementari che spettano ad ogni persona, che siano considerati, questi, non solo come una conseguenza della ripresa dei negoziati politici, ma come un qualcosa che ha valore in sé, indipendente, che non può essere subordinato agli sviluppi della stessa vicenda nella quale, certo, tale questione è inserita. Per questo vogliamo chiedere di nuovo che osservatori internazionali possano vedere Gilad Shalit, che la Croce Rossa possa verificare le sue condizioni di salute, che siano, in altre parole, rispettati i suoi diritti.

dall'anonimato delle statistiche comunicate dagli opposti Stati maggiori, di statistiche che ci consegnano una situazione in cui i nomi ed i volti spariscono. Forse cercare di ritrovare i lineamenti di un volto ed ascoltare la trepidazione nelle parole e negli sguardi di un padre è qualcosa

Ho visto un uomo che interpreta la lotta per la vita di suo figlio e per la difesa della sua famiglia come una lotta per valori universali. Un uomo dalle cui parole e gesti è estraneo l'odio ed è portatore di un profondo messaggio di amore. Per questo credo che l'approvazione di questa mozione sia anche un omaggio ad un uomo riuscito, in questa drammatica ed incredibile circostanza, ad interpretare in questo modo il suo ruolo e la sua opposizione.

Signora Presidente, colleghi senatori, la vicenda di questo giovane caporale israeliano, Gilad Shalit, è emblematica della drammatica situazione in cui versa la tutela dei diritti umani e delle libertà dell'individuo nell'ambito del conflitto israeliano-palestinese. Gilad non aveva vent'anni, aveva da poco dato l'esame di maturità e da soli undici mesi prestava il servizio militare obbligatorio quando, il 25 giugno 2006, fu rapito. Ne compirà 23 il prossimo 28 agosto. Sono infatti trascorsi tre lunghi anni da quando fu sequestrato da terroristi da Hamas, che fecero irruzione sbucando da un tunnel sotterraneo a Kerem Shalom, in territorio israeliano, uccidendo due soldati israeliani e ferendone altri quattro. Impossibile non condannare questo atto efferato, assolutamente ingiustificabile. Vale la pena, infatti, ricordare che all'epoca del rapimento Gaza era già stata totalmente evacuata sia dall'esercito israeliano che dai coloni ebraici. giorni dopo il rapimento di Gilad, dal Libano meridionale, anche in questo caso territorio libero e sovrano interamente evacuato dall'esercito israeliano, un commando di terroristi libanesi sciiti dell'Hezbollah si spinsero in territorio israeliano e rapirono due soldati. I loro corpi sono stati restituiti il 16 luglio 2008 in cambio di terroristi detenuti nelle carceri israeliane. Invece Gilad, ad oggi, è ancora prigioniero, nonostante la mediazione egiziana condotta nell'ambito del rilascio di alcuni prigionieri israeliani. Né se ne conoscono le condizioni psicofisiche. Infatti, da tre anni a questa parte nessuno lo ha potuto visitare, neppure il padre. Anche la Croce Rossa internazionale è tenuta lontano. Questa situazione contravviene con qualsiasi convenzione internazionale a tutela dei diritti umani e in particolare dei prigionieri. Di fronte all'indifferenza e al silenzio assordante dell'Europa, plaudiamo quindi all'iniziativa italiana, promossa dalla Commissione per i diritti umani, che nel corso di una recente missione a Gaza, in Cisgiordania e in Israele, incontrando, fra gli altri, gli esponenti della comunità italiana in Israele, presieduta da Beniamino Lazar, ha accolto l'invito a seguire la drammatica vicenda del caporale Shalit. L'attenzione del Parlamento su questa vicenda ha incontrato la sensibilità del Comune di Roma. Oggi Shalit è cittadino italiano, avendo ricevuto in Campidoglio la cittadinanza onoraria, alla presenza del padre, udito il 1° luglio in Commissione diritti umani. È un cittadino onorario italiano prigioniero, per questo l'impegno del nostro Paese è di primaria importanza. è anche un cittadino onorario dell'Europa, è quindi auspicabile un impegno per la sua liberazione anche da parte europea. Una liberazione che non solo dovrebbe risolversi in uno "scambio di prigionieri", quale risarcimento morale per le sofferenze patite da entrambi i popoli, ma soprattutto una liberazione che dovrebbe collocarsi nel solco di un reciproco impegno alla promozione e tutela dei diritti umani nell'ambito del conflitto israeliano-palestinese, a difesa della sacralità della vita e delle libertà fondamentali e per la ripresa del processo di pacificazione. Nel sostenere quindi la politica sino ad oggi condotta dall'Italia affinché il processo di pace riprenda, nel riconoscimento reciproco dei diritti del popolo israeliano e di quello palestinese e nel reciproco riconoscimento dei due Stati, preannuncio il voto favorevole del mio Gruppo

è giustissimo l'impegno della Commissione diritti umani del Senato per la liberazione di questo soldato israeliano prigioniero

notizie, questo ci obbliga a prendere sul serio la preoccupante asimmetria della situazione esistente nei territori palestinesi, testimoniata da tutti gli organi internazionali d'indagine,

di così impressionante disparità nel numero delle vittime e nei dati riferiti al danno inferto alle popolazioni, da farci rimanere disarmati di fronte alla possibilità di una risoluzione positiva.

dalla lotta per il possesso di una sola terra. È giusto che, sia nella risoluzione del Parlamento

per così dire - dell'intelligencija israeliana, grandi scrittori che tutti siamo abituati a leggere, anche per diletto,

Dall'interno stesso dell'opinione pubblica israeliana vi è una pressione a fare in modo che la risoluzione di questo conflitto passi attraverso un accordo sulla divisione consensuale delle terre e sul riconoscimento reciproco.

la fiamma del conflitto. Lo stesso evento da cui nasce questa vicenda ne è un esempio: in una situazione di parziale allentamento delle ostilità, è bastato un singolo atto di guerra per riavviare tutta la logica e riportare la vicenda nella dimensione di uno scontro fragoroso e generale, che sfascia le città, uccide le famiglie, nega il diritto al nutrimento e all'istruzione. Che dire? Si è incapaci di proporre una soluzione. Tuttavia, pur nella sensazione precisa e disarmante di questa incapacità, abbiamo sentito la necessità di firmare questa mozione, con la convinzione più convinta: non c'è altro da fare che portare il proprio granello di sabbia, uno dietro l'altro. Questo non sarà l'ultimo, ma dovremo continuare a farlo.

circostanze offrano quelli che, con espressione confacente, vengono definiti momenti alti della vita istituzionale. Frangenti in cui, al cospetto di drammi collettivi e personali, l'azione politica dà prova di non ridursi all'*hortus* *conclusus* dei riti di Palazzo e invece si fa carico delle tribolazioni dei popoli o dei singoli rendendosi portatrice della speranza che nasce dalla solidarietà e dall'impegno. In tale contesto, la vicenda del signor Noam Shalit acquista una prospettiva che va oltre la sofferenza del padre a cui è stato strappato il figlio, soldato ventenne, per inserirsi nel più ampio scenario di quelle battaglie di progresso civile che abbracciano l'intero genere umano. Appare di scarso rilievo che il caporale Gilad Shalit, detenuto da oltre tre anni in una prigione di Hamas, militi nei ranghi delle Forze armate israeliane, come risulta del tutto trascurabile conoscerne il credo religioso: dei diritti umani, con il proprio documento, riafferma il principio di valore universale per cui nessuna persona, per alcuna ragione al mondo, può essere privata dei diritti che le Convenzioni internazionali riconoscono ai detenuti e ai prigionieri. Mi rendo conto del rischio di cadere nella vuota enunciazione, per come questa affermazione viene smentita dalle prassi quotidiane di soprusi e violenze, orrori che certo non risparmiano lo scenario mediorientale in cui si sta consumando il dramma del caporale Shalit tuttavia, colleghi senatori, un Parlamento e un Governo che considerano la centralità della dignità umana come pietra miliare di civiltà evidentemente posseggono molti strumenti in più del genitore che si batte perché in nome di questi stessi valori gli sia reso un figlio. Dunque non possiamo - e certo non intendiamo - sottrarci a tanta sfida, ad una prova che va affrontata con le armi lungimiranti della politica, trascendendo la vicenda personale e collocandola in un contesto più generale che reclama soluzioni. In questo senso, la mozione della Commissione conviene che la liberazione del militare israeliano rappresenti «un tassello fondamentale per la ripresa del processo di pace interrotto». Così, mentre si impegna il Governo a promuovere ogni possibile azione perché Gilad Shalit venga liberato, si ribadisce l'urgenza di quel processo di pace che deve riprendere dall'assunto dei «due popoli, due Stati» e dal riconoscimento reciproco delle sofferenze patite da ambo le parti in tanti anni di conflitto dagli elevatissimi costi umani. Certamente costituiscono motivo di particolare afflizione le ostilità feroci che contrappongono nell'odio e nel sangue versato popolazioni che condividono la stessa terra e persino l'identico ceppo. Dolorosamente e con il dovuto riguardo per i tragici scenari che questa espressione evoca, si potrebbe parlare dello scandalo di un reciproco antisemitismo: potremmo esprimerci in questi termini considerando quali e quanti siano i fattori che legano ebrei e palestinesi, in una contiguità che va ben oltre l'attuale convivenza forzata e che si sostanzia nella medesima appartenenza semitica. attribuzione di semitismo testimonia la Bibbia, precisamente nel capitolo della Genesi, ove vengono elencate le Nazioni che compongono la discendenza di Sem, figlio del patriarca Noè. Ricordo anche come l'analoga definizione assimili questi due popoli secondo il criterio vigente in campo linguistico per classificare le popolazioni di idioma semitico.

dalle correlazioni del cromosoma Y hanno dedotto la seria possibilità di una comune ascendenza di ebrei e palestinesi. Non per nulla, studiosi israeliani - ultimo nell'ordine di tempo è il clamoroso caso di Shlomo Zand, autore di un *best seller*

si sono spinti sino a sostenere che i palestinesi siano i discendenti di quella parte dell'antica popolazione ebraica che evitò la diaspora, rimase nella propria terra e finì per convertirsi all'Islam in seguito all'espansione maomettana. argomentazioni dovrebbero indurci a riflettere non meno delle quotidiane sofferenze sulla tragica assurdità del conflitto israelo-palestinese. Così, il caso umano portato alla nostra attenzione ci induce a riconoscere, negli occhi di un genitore, l'immagine del dolore delle persone troppo spesso oscurata dalla retorica nazionalista e dalla propaganda di parte. A un giornalista che gli chiede quanto sia difficile il ruolo di padre e patriota, il signor Noam Shalit in maniera disarmante risponde: «Non sono un patriota, sono solo un padre». Credo che il nostro Governo potrà sollecitare la liberazione del prigioniero esprimendosi a nome del diritto violato, ma anche delle resistenze calpestate visto che, a fronte del riconoscimento politico preteso da Hamas, questa mozione domanda ai contendenti il reciproco riconoscimento delle sofferenze causate indiscriminatamente. Forse per la prima volta un documento politico afferma che l'angoscia e il dolore di chi non può più riabbracciare la persona cara non costituiscono un fatto accidentale della crisi israelo-palestinese come, peraltro, di qualsiasi conflitto. Posta in questi termini, con una premessa di autentica umanità fatta propria da ambo le parti, la pur doverosa e auspicata liberazione di Gilad Shalit costituirebbe una svolta politica senza precedenti. Tra ebrei e palestinesi sinora hanno prevalso le trattative imbastite per strappare qualche vantaggio a discapito del contendente; otterremmo invece un risultato di inestimabile valore se, in virtù della missione di un padre e dell'impegno di quanto l'hanno sostenuto,

a parlarci di suo figlio prima di andare a Ginevra per deporre davanti alla Commissione delle Nazioni Unite per volere dell'Alto commissario per i diritti umani delegato, su mandato del Consiglio delle Nazioni Unite per i diritti umani, a

questioni che hanno a che fare sicuramente con un dramma umano, che speriamo non evolva in tragedia, altrettanto sicuramente con la cogenza del diritto internazionale e, infine, con la situazione politica generale che attiene alla pace in Medio Oriente.

di sanzioni a livello internazionale per quanto riguarda il diritto consuetudinario. È noto, infatti, che Israele e l'Autorità nazionale palestinese, che comunque non rappresenta ancora e poi ci arriveremo - uno Stato indipendente, riconoscono la giurisdizione dell'altro organo permanente che avrebbe competenza per giudicare i crimini internazionali, vale a dire la Corte penale internazionale, davanti alla quale però i palestinesi vorrebbero che Israele venisse portato per il modo in cui il conflitto, dall'inizio dell'anno, è stato condotto dall'esercito israeliano. Noam Shalit, il padre di Gilad, dopo aver raccontato a noi che cosa sta vivendo da tre anni a questa parte, ha deposto davanti alla Commissione delle Nazioni Unite, presieduta dal giudice Goldstone, che dovrebbe

rapito un figlio di cui non si hanno notizie, salvo una breve videocassetta in cui si riesce a capire che in effetti Gilad è ancora vivo.

e perché il processo di pace possa riprendere dall'assunto "due popoli, due Stati" e dal riconoscimento reciproco delle sofferenze patite da ambo le parti in tanti anni di conflitto e dagli elevatissimi costi umani».

causa anche il ruolo che l'Iran direttamente ed indirettamente, attraverso la Siria e i suoi tentacoli in Libano, ha giocato nella destabilizzazione permanente della regione.

magari era felice nel momento in cui è stato pronunciato la prima volta (perché due popoli che hanno dimostrato ampiamente di non voler vivere insieme non devono vivere insieme), fino ad allora la pace non sarà alla nostra portata. La pace oggi sarebbe soltanto fotografare l'esistente. Ammesso e non concesso che comunque i soggetti da coinvolgere non sarebbero soltanto il Governo israeliano, ma anche due fazioni palestinesi spesso in conflitto fra di loro, riprenderebbe uno Stato democratico che, in virtù della necessità di affermare la propria sicurezza spesso arriva a sospendere - ahinoi - molte delle libertà civili che, comunque, continuano a caratterizzarlo come l'unica democrazia in Medio Oriente (ancora di più della Repubblica turca).

se diventeranno una democrazia potranno avere la speranza di vedere i principi di libertà, giustizia e Stato di diritto garantiti per i milioni di israeliani e per i milioni dai palestinesi. Quindi, recuperando uno *slogan* efficace ma - ahinoi - non praticato in buona fede dell'Amministrazione Bush, occorre sperare che un effetto domino possa interessare tutti i Paesi che circondano questo territorio: laddove la democrazia è debole e fragile, come in Libano e in Giordania, e laddove stenta a manifestarsi nei suoi tratti liberali, come in Egitto. Il Congresso del 2008 dei Radicali Italiani ha adottato una raccomandazione nella quale si invitavano i parlamentari radicali italiani ed europei a promuovere una missione parlamentare a Gaza, che si impegnasse a non lasciare la Striscia fino a quando non si sarebbe potuto incontrare il soldato Shalit e verificare le sue condizioni di salute. La missione avrebbe dovuto essere di carattere umanitario, aperta a chiunque intendesse parteciparvi e, se necessario, i gruppi di parlamentari di tutti gli schieramenti politici avrebbero dovuto garantire una loro presenza *in loco* fino al giorno in cui Gilad Shalit non fosse stato liberato da Hamas. Non abbiamo trovato la forza (ma per certi aspetti forse bisognerebbe chiamare in causa anche il coraggio) di andare a Gaza e imporre questo, perché sarebbe stata forse una delle classiche

Signora Presidente, il collega Marcenaro ha ricordato, con molta precisione e con molta eleganza, il senso dell'incontro che due settimane fa molti di noi, grazie alla Presidenza del Senato, hanno potuto avere con il padre di Gilad Shalit. Ecco, quello del padre è un argomento risuonato nella nostra discussione. Soprattutto un padre, anzi soltanto un padre, non un patriota e non un uomo politico, perché lo Stato di diritto e la democrazia non hanno il diritto di chiedere a un padre di essere anche un patriota. Da questo punto di vista, la vicenda esalta le ragioni che fanno di Israele, unico nella Regione, uno Stato di diritto e una democrazia. Ovviamente l'altra faccia del problema è Gilad Shalit è un soldato delle Forze armate israeliane; queste sono esercito di popolo, nell'accezione più democratica e mazziniana del termine. Di qui quel patto che impone allo Stato di fare di tutto per salvare le vite umane e, dopo aver fatto di tutto per salvare le vite umane, fare ancora di più per recuperare i corpi. Di qui la ricattabilità dello Stato di Israele in questa vicenda. I miei sentimenti politici sono ovviamente più vicini a quelli del senatore Perduca che a quelli del senatore Pardi sulla valutazione di interlocutori come Hamas e Hezbollah, ma soprattutto la mia ricostruzione della vicenda è quella del collega Perduca, anche nelle implicazioni di diritto internazionale.

una collega che ha la Croce Rossa nel cuore, assai più di me. La conobbi al principio degli anni '90 - lei era giovane sottosegretaria al Ministero della sanità - proprio per vicende riguardanti la Croce Rossa.

ma il punto veramente sconvolgente è che in tre anni la Croce Rossa internazionale brilla per inerzia, cioè per opacità e - se mi è consentita molta franchezza - per viltà. È una viltà inaccettabile il fatto che la Croce Rossa internazionale, attivissima da sempre nella Striscia di Gaza, in questi tre anni non risulta essersi mossa

c'è una lettera di Gilad un mese dopo, alla fine di luglio, fatta pervenire non attraverso la Croce Rossa, ma attraverso dei benemeriti mediatori egiziani (primo momento di opacità o, meglio, di viltà); un anno dopo c'è il video con Shalit che parla con voce provata; il terzo - siamo al giugno 2008 - una lettera alla famiglia. Nulla è passato per la Croce Rossa internazionale. Questa Croce Rossa si muove dentro la Striscia di Gaza,

non già dell'esercito israeliano, ma collaborazionisti palestinesi con altri palestinesi; questa Croce Rossa, all'indomani della vicenda bellica del gennaio scorso, ha accusato l'esercito di Israele, infangando l'onore dei suoi ufficiali e dei suoi soldati, di non

Mi domando allora come sia possibile che la Croce Rossa internazionale abbia aggirato completamente la vicenda alla quale nobilmente il Gruppo del PdL aderisce. Il collega Marcenaro dice di aver presentato una mozione perché l'odiosità, la ricattabilità sul corpo, sulla vita dei figli con i padri deve pur avere un limite,

non ha mai voluto accogliere in seno alla propria organizzazione la Stella di David Rossa, la quale ha il merito, a trecentosessanta gradi, di essere sempre pronta a correre nel mondo dove c'è una calamità. La Croce Rossa internazionale non l'ha voluta, perché la Stella di Davide è un fatto religioso, mentre invece accoglie pienamente e collabora, proprio nei territori della Striscia di Gaza, con quella Mezzaluna Rossa la quale, invece, esclude la possibilità di prestare soccorso a cristiani, ebrei e credenti in altre religioni. Da questo punto di vista avremmo voluto che da parte degli organi della comunità internazionale, in nome delle norme evocate dal senatore Perduca

a far piangere le stesse lacrime ad Achille e a Priamo, fosse stato messo al centro dell'attenzione questo imperdonabile, inescusabile ruolo della Croce Rossa internazionale.

l'antisionismo è solcato da molto antisemitismo, come dimostra la ridicola commedia della Federazione internazionale della stampa che, più o meno con gli stessi argomenti poi negati dalla Croce Rossa internazionale, si permette di comminare l'espulsione dei giornalisti israeliani dalla Federazione. L'ultima notizia, di oggi, riporta che non hanno pagato le quote;

Comunque, rimandando ad altra occasione il dibattito politico su Hamas, Hezbollah e tutt'altro, i sentimenti e gli argomenti per i quali il collega Marcenaro ha

ha alcuna giustificazione militare e rappresenta un ricatto inaccettabile non solo per il Governo d'Israele, ma per tutta la comunità internazionale. L'Italia sostiene le ragioni del signor Shalit e si è unita in numerose occasioni agli appelli da lui lanciati per la liberazione del figlio e la fine di quel regime oppressivo ed estremista che condanna la popolazione della striscia di Gaza. Il Ministro degli affari esteri è sempre stato vicino alla famiglia del soldato rapito, che ha incontrato durante la sua ultima visita compiuta in Israele lo scorso 20 gennaio, all'indomani della conclusione - grazie anche all'intensa azione diplomatica sviluppata dall'Italia - del conflitto nella striscia di Gaza. Nuovamente il Ministro degli esteri e il signor Shalit si sono incontrati, proprio qui, nelle Aule del Senato, lo scorso 1° luglio. Questo nuovo incontro ha consentito di rinnovare da parte del Governo italiano il rispetto e la vicinanza al dramma che la famiglia sta vivendo e di condividere pienamente anche l'alto significato morale della concessione della cittadinanza onoraria da parte del Comune di Roma. Gli sviluppi della situazione sul terreno lasciano periodicamente sperare e pensare che il rilancio dei negoziati per la liberazione del giovane possa avvenire anche tramite la scarcerazione di altri detenuti palestinesi richiesta da Hamas. Il Governo italiano monitorizza e segue costantemente la situazione, comprendendo come questo alternarsi di notizie e di speranze sia particolarmente doloroso per la famiglia. L'Egitto - com'è noto - sta conducendo una delicata e discreta azione di mediazione, che l'Italia non cessa di sostenere assieme a tutti i Paesi della Comunità Europea. In questo contesto, anche nel quadro della Presidenza del G8, l'Italia è in prima linea nel promuovere una ripresa senza condizioni dei negoziati che porti rapidamente, in un quadro più generale, anche ad una soluzione giusta del conflitto mediorientale, basato sul principio dei due Stati e sulla creazione di uno Stato palestinese indipendente, democratico, vitale e contiguo, che viva in pace con tutti i suoi vicini, nel riconoscimento dei confini e della sicurezza dello Stato di Israele. Pertanto, il Governo esprime parere favorevole sulla mozione n. 150, presentata

Signora Presidente, il Gruppo del Partito Democratico voterà, con convinzione, a favore di questa mozione che vede come primo firmatario il senatore Marcenaro, presidente della Commissione per la tutela e la promozione dei diritti umani, e che è sottoscritta dai colleghi di tutti i Gruppi. Nella mozione si chiede al Governo di adoperarsi con il massimo sforzo per avvicinare la liberazione del giovane soldato israeliano Gilad Shalit frattempo di consentire l'ottenimento di informazioni circa le sue condizioni di prigionia e il suo stato di salute. Com'è stato ricordato, Gilad Shalit non è un prigioniero di guerra, perché è stato sequestrato mentre pattugliava il territorio del suo Paese da tre anni - noi tutti speriamo che viva - senza che nessuno della sua famiglia e nessun organismo umanitario abbia potuto visitarlo e verificare il suo Il dramma suo e della sua famiglia parlano certamente di una violazione inaccettabile dei diritti umani fondamentali, ma credo che parlino anche molto di politica. Parlano, con tragica evidenza, delle ragioni più profonde che hanno impedito finora di trovare una soluzione alla guerra, più o meno strisciante e dichiarata, che oppone da decenni Israele ai Paesi arabi, Israele ai palestinesi. Alla radice del rapimento di Gilad c'è lo stesso grumo di odio che ha impedito finora di mettere la parola fine al conflitto israelo-palestinese nell'unico modo legittimo e realistico, quello dei due popoli-due Stati. C'è la negazione dell'altro, la negazione della sua umanità anche come nemico. Questo immenso ostacolo alla pace non si vede all'opera, dobbiamo dirlo, soltanto nella vicenda di Gilad Shalit. Per esempio, cito qualcosa che ho visto con i miei occhi poche settimane fa visitando la Cisgiordania con una delegazione della Commissione per i diritti umani, la stessa negazione dell'altro si vede nell'odio quasi atavico che spinge a Hebron i bambini israeliani, figli dei coloni, a gettare rifiuti ed escrementi sulle vie del suk. Aggiungo, non per polemizzare con nessuno ma per amore di verità, che la negazione dell'altro trova alimento anche nelle timidezze, nelle ambiguità di organizzazioni e movimenti che di fronte alla tragedia mediorientale sembrano mossi da una capacità di indignazione selettiva, che è indeflettibile quando ci sono da condannare la rigidità e le ingiustizie che vedono come imputato Israele e che invece è assai più elastica, talvolta molto distratta, se c'è da censurare con forza comportamenti e posizioni inaccettabili da parte palestinese. Per esempio, come è stato ricordato, in questi anni, proprio nel caso di Gilad Shalit non si è sentita la voce dei movimenti pacifisti e abbastanza flebile e discontinua è stata la stessa voce di autorevolissimi organismi umanitari internazionali. Riconoscere l'altro, anche quando veste i panni del nemico, questa è la sola via d'uscita dall'inferno mediorientale. È la via battuta in passato da grandi uomini come Yzak Rabin, è la via che fece dire a Moshe Dayan, l'eroe della Guerra dei sei giorni, che per fare la pace si deve parlare con i nemici, non con gli amici. È la via indicata oggi, con passione e sofferenza, da altri grandi uomini come David Grossman, che invita gli israeliani a guardare con gli occhi del nemico. Questa è anche la via scelta da Noam Shalit, padre di Gilad, nel suo pellegrinaggio instancabile per avvicinare il giorno della liberazione di suo figlio. Noam Shalit non ha risposto con l'odio all'odio cieco e disumano di cui è vittima; anzi, ha fatto di se stesso un messaggero di dialogo e anche nel dolore terribile di questi tre anni si è sempre sforzato di guardare con gli occhi del nemico. Anche Gilad è una persona che ha sempre voluto guardare con gli occhi del nemico. Non ho ora il tempo di leggerla, ma invito tutti voi a leggere una brevissima favola che Gilad Shalit scrisse quando aveva 11 anni, e che ora è pubblicata anche in Italia per iniziativa dell'associazione che porta il suo nome. La favola si intitola «Lo squalo e il pesciolino» e racconta di uno squalo che incontra un pesciolino e invece di mangiarlo ci fa amicizia.

Noi che per nostra fortuna viviamo in un Paese che è in pace non possiamo probabilmente erigerci a giudici delle ragioni e dei torti di israeliani e palestinesi, ma dobbiamo aiutare gli uni e gli altri a trovare in se stessi la forza di un umanesimo che si faccia più forte della negazione dell'altro, un umanesimo senza il quale questa moderna terribile guerra dei cent'anni non finirà. La mozione che ci accingiamo a votare è un piccolo, ma io credo prezioso, contributo in questa direzione, come lo è stato il conferimento a Gilad Shalit della cittadinanza onoraria di Roma decisa dal sindaco Alemanno: Gilad oggi è anche nostro concittadino. In qualche modo io auguro a lui, auguro a me stesso e auguro a tutti noi di poterlo presto ospitare in Italia, anche in Senato, come uomo finalmente libero e come testimone di pace

giungendo a pretermettere - dice qualcuno fondatamente - i propri diritti e le proprie richieste motivate,

la Repubblica di Slovenia ha posto barriere piuttosto forti, talché ad oggi, nonostante la Croazia abbia oggettivamente fatto progressi significativi purtroppo - grazie o a causa della posizione della Repubblica di Slovenia - non si è riusciti ancora (e si teme per parecchio tempo non si riuscirà) a definire l'ingresso della Croazia nell'Unione europea. Qual è la situazione delineata nella nostra mozione? Innanzitutto, si parla del permanere delle attese degli esuli italiani di Istria, Fiume e Dalmazia. Questo che risale al dopoguerra

quanto specificamente legato alla restituzione degli immobili ancora restituibili in quanto nazionalizzati; al riguardo (mi riferisco alla Croazia, posto che a tale riguardo non vi sono state aperture da parte della Slovenia),

la guerra, il dopoguerra, il regime dittatoriale della Jugoslavia e tutte le situazioni che storicamente conosciamo), hanno dovuto abbandonare i territori assegnati alla ex Jugoslavia; e di questo ho fatto cenno;

un significato storico);

un *agreement,* un accordo tra Italia e Croazia per cui tanti soldi vengono dati dall'Italia alla minoranza italiana italiana in Croazia ed altrettanti vengono dallo Stato croato. Nell'ultima finanziaria circa un terzo di tali fondi, peraltro modesti, sono stati tagliati. Quindi, bisogna

si addivenga ad una qualche forma di sistema finanziario agevolato per l'acquisto, in particolare degli esuli istriani, giuliani e dalmati, di beni che si trovino nella Repubblica croata e, aggiungo, nella Repubblica slovena, magari istituendo fondi di garanzia gestiti da banche nazionali italiane.

a mio avviso, l'esame del documento alla nostra attenzione consente di svolgere, seppure in modo parziale, una comune riflessione su un argomento particolarmente delicato e significativo qual è il processo di stabilizzazione dell'Europa centrale e balcanica. tema di particolare interesse, soprattutto per alcune zone del nostro territorio nazionale che, per ragioni storiche, culturali ed economiche, mantengono da tempo stretti rapporti con le popolazioni che in quell'area risiedono e alle quali sono legate per avere vissuto in comune tanta parte della loro storia. Infatti, il processo avviato per l'ingresso a pieno titolo nell'Unione europea della Croazia rappresenterà, una volta conclusosi (ed io credo positivamente), un tassello fondamentale nel consolidamento della stessa Unione europea. si andrà configurando la realizzazione in quell'area così delicata dell'Europa di un ulteriore passo in avanti rispetto ai processi di disgregazione a forte impronta nazionalistica, che hanno caratterizzato la vita di quei Paesi e di quelle popolazioni anche nel più recente passato. Per il Governo di Zagabria il rapporto con il nostro Paese è un punto fondamentale del suo cammino verso l'integrazione europea. In tale quadro, vanno segnalati alcuni importanti aspetti dei rapporti bilaterali fra l'Italia e la Croazia. Le relazioni fra i due Paesi sono da tempo forti e intense in ogni settore, al punto che l'Italia è oggi il primo partner commerciale della Croazia. Si tratta di relazioni costruite nel corso di un quindicennio da tutti i Governi che si sono succeduti alla guida del nostro Paese Paese e che hanno consentito di cominciare a sanare con coraggio vecchie incrostazioni e di avviare il superamento di problemi che parevano irrisolvibili. Fra questi vi è indubbiamente il tema dell'annoso negoziato sui beni degli esuli e le difficoltà di collaborazione nei settori marittimo, ambientale e delle risorse ittiche in Adriatico. Va in ogni caso positivamente segnalato il fatto che, fra le questioni ancora aperte, risulta superato in via formale il tema dell'accesso al mercato immobiliare croato e delle discriminazioni cui erano di fatto sottoposti i cittadini italiani. Questi positivi rapporti bilaterali sono, quindi, un aspetto di grande utilità nell'avvicinamento della Croazia all'Unione europea e per la sua, più rapida possibile, integrazione. Da più parti viene sottolineato che il 2009 sarà l'anno decisivo per una buona soluzione del negoziato europeo. Nell'ambito dei punti posti al centro del negoziato, molte questioni sono state risolte, pur permanendo, come è noto, un difficile contenzioso sulla questione delle acque territoriali con la Repubblica di Slovenia. A ciò si aggiunge ora, purtroppo, una difficile fase politica della Croazia, recentemente sfociata nelle dimissioni del primo ministro Ivo Sanader e nella nomina del nuovo Governo guidato da Jadranka Kosor. Il difficile momento politico della Croazia si accompagna, inoltre alla crisi economica, che sta investendo anche Zagabria come gli altri Paesi dell'area balcanica. In ogni caso, va tenuto presente che l'attuale Governo di centrodestra guidato dall'HDZ, così come l'opposizione di centrosinistra, sono concordi nel perseguire la strada dell'integrazione europea. Come detto, anche nel nostro Paese maggioranza e opposizione sostengono il percorso croato di adesione quale elemento centrale dei processo di stabilizzazione e di progresso dell'intera area balcanica. In questo, vi è la comune consapevolezza che il processo di integrazione della Croazia nell'Unione europea comporterà sicuramente anche il superamento delle questioni bilaterali ancora aperte e porrà in essere il pieno rispetto delle minoranze linguistiche, così come un elevato standard di diritti civili. Infatti, il processo di adesione risulta un passo significativo, in particolare per i circa 30.000 cittadini croati di lingua italiana. A tal proposito, voglio far osservare all'Aula, a testimonianza dei profondi legami che uniscono questi cittadini croati di lingua italiana al nostro Paese, che ben 9.000 di essi sono iscritti nell'apposito registro AIRE della città di Trieste; è quindi evidente il loro interesse e legame alla vita istituzionale, politica e sociale del nostro Paese. Si tratta, dunque, signora Presidente, in questa fase delicata e decisiva del processo di integrazione, di seguire con attenzione, usando tutti gli strumenti diplomatici che abbiamo a disposizione, gli interessi della minoranza italiana in Croazia. Ciò va fatto non solo per affermare ogni tutela prevista agli italiani lì residenti, ma anche per costruire le dovute risposte alle annose richieste e speranze di coloro i quali abbandonarono l'Istria, Fiume e la Dalmazia e che da troppo tempo - lo sottolineo - chiedono la salvaguardia dei loro diritti. In tale contesto va in ogni caso ribadita, a supporto dei contenuti della mozione, la necessaria prosecuzione del lavoro avviato nel tavolo Governo-esuli, per determinare tutte le condizioni utili al possibile indennizzo e restituzione dei beni espropriati nell'immediato dopoguerra. In conclusione, a mio avviso, è necessario che il Governo italiano mantenga viva e forte la sua azione in questa fase decisiva dell'adesione della Croazia all'Unione europea, affinché i diritti degli italiani che vi risiedono siano pienamente tutelati e perché si giunga a risolvere positivamente la questione dei beni espropriati agli esuli. In tal modo potremo, noi tutti insieme, scrivere una pagina importante nella storia del nostro continente, dando così ulteriore impulso alla costruzione di una forte ed estesa soggettività politica dell'Unione europea.

che l'aveva liberata dall'occupazione nazista grazie allo sforzo congiunto della resistenza locale, sia slava che italiana. Tuttavia, la politica di persecuzioni, vessazioni ed espropri messa in atto da Tito ai danni degli italiani, culminata nel dramma delle foibe, già sperimentata nel settembre del 1943, spinse la massima parte della popolazione locale di etnia italiana ad abbandonare l'Istria, dando vita ad un vero e proprio esodo.

legato a radici storiche di un problema che il nostro Paese da tempo si trova a dover affrontare nell'area istriana, fiumana e dalmata. Per lunghi anni ci siamo trovati a negoziare su tale problema, sulla questione del risarcimento dei cittadini italiani che hanno dovuto lasciare la loro terra natale tra il 1945 e il 1954, i cui beni, come sappiamo, vennero espropriati da Tito. Accanto al problema dei profughi, vi è inoltre quello dei pochi italiani che scelsero di restare in Istria e in Dalmazia, una minoranza linguistica ancora oggi discriminata, anche se meno di un tempo. Un esempio è quello riportato dalle Associazioni degli esuli giuliano-dalmati che più volte, infatti, hanno ribadito la loro posizione sul delicato ed urgente tema dei documenti di identità e dei codici fiscali, dal quale - cito - «discendono umilianti ed inaccettabili disagi per gli esuli in tutte le sedi amministrative, dai ricoveri ospedalieri alle operazioni bancarie». Oggi la Croazia si sta avviando verso l'Unione europea ed è questa un'opportunità eccellente per chiedere al Governo italiano di riaprire per l'ennesima volta il negoziato, esercitando ogni pressione lecita sulla Croazia, affinché venga applicata la stessa legge che Zagabria applica ai cittadini croati, senza discriminazioni, che la normativa comunitaria non tollera. Ricordo che la Croazia, dopo aver presentato domanda nel 2003 per l'ingresso nell'Unione europea, nel 2004 è diventata ufficialmente candidato dell'Unione. I negoziati avviati dal Consiglio dell'Unione europea dovrebbero verosimilmente portare la Croazia nell'Unione entro

ragion per cui ci sembra il momento più opportuno per chiedere al Governo di impegnarsi in maniera incisiva a favore di quella minoranza italiana (circa 30.000 cittadini) ancora in attesa di veder rispettati i propri diritti. La Croazia, a dire il vero, ha finora dimostrato scarsa disponibilità nel dare risposte concrete al problema della restituzione dei beni a suo tempo espropriati dall'ex regime comunista di Tito ai cittadini italiani che Vorremmo quindi che, prima che il Parlamento italiano desse il via definitivo all'adesione della Croazia all'Unione europea, la trattativa bilaterale attualmente in corso per la restituzione dei beni degli esuli italiani fosse conclusa o raggiungesse qualche risultato favorevole.

e che pure ha dovuto affrontare il problema della minoranza dei cittadini tedeschi e soprattutto dei cittadini che hanno dovuto lasciare la loro terra,

Questa minoranza tedesca è stata risarcita, anche se a dire la verità non in modo completamente soddisfacente, soddisfacente, dalla Repubblica Ceca prima che essa entrasse a far parte della Comunità europea, come si chiede che venga fatto oggi dalla Croazia. Per i motivi fin qui quindi esposti, sosteniamo questa mozione,

a lavorare per il pieno rispetto degli accordi italo-croati a tutela della comunità nazionale italiana residente nella Repubblica di Croazia, nel quadro della normativa comunitaria

competenti organi comunitari, con particolare riferimento alla tutela delle minoranze ed in particolare della minoranza italiana, possa celermente entrare a pieno titolo nell'Unione europea. Signora Presidente,

Dopo la Seconda guerra mondiale, il Sudtirolo ha visto svanire le proprie speranze di autodeterminazione proprio per il distacco dell'Istria dall'Italia: l'Italia, dopo aver perduto l'Istria, Fiume e Zara rischiato addirittura di perdere Trieste e Gorizia, non voleva e forse non poteva rinunciare al Tirolo del Sud. È pertanto per noi un'occasione preziosa, come minoranze oltre che come cittadini di questo Paese e dell'Europa,

includendo argomenti di carattere più generale che vanno anche oltre l'oggetto delle stesse, e mi pare che l'ultimo intervento abbia abbondantemente dato prova di questo, anche se, fortunatamente, non è scritto nella mozione. Faccio mie tutte le considerazione del senatore Pegorer, articolate poco fa a nome del Gruppo del Partito Democratico, spiegando perché mi sono iscritto a parlare Il quarto impegno che si chiede al Governo con questa mozione è, "nel quadro della normativa comunitaria sul rispetto delle minoranze e nello spirito di un'integrazione di regioni la cui fisionomia nazionalismi e totalitarismi hanno devastato nel '900", di tutelare i diritti di una minoranza.

dell'ex Stato della Federazione jugoslava che invece si trovano in Italia. Noi ci troviamo oggi ad affrontare un documento con cui la maggioranza ha sollevato un problema (salvo poi non essere presente in forze al dibattito di oggi), su cui il Governo probabilmente darà un parere favorevole, salvo poi non mandare i rappresentanti del Ministero che si dovranno interessare di questo, e a fare dei ragionamenti che fortunatamente, grazie al negoziato che si è svolto preventivamente nella preparazione di questo documento, hanno incluso il tema nel perimetro delle istituzioni europee,

auspicata qui dentro, ma anche a quella necessaria per arrivare a risolvere il problema grazie alle norme europee che ci siamo dati negli ultimi quattro decenni. Si tratta, quindi, di questioni di regioni e di minoranze. proprio per dare il messaggio agli italiani e anche agli altri europei che ci sono degli italiani che si interessano sia delle minoranze italiane all'estero che delle minoranze straniere in Italia (cosa che questo Governo gestisce molto spesso attraverso il codice penale piuttosto che con politiche sociali sociali o di tipo diverso), ho deciso con la senatrice Poretti di presentare un disegno di legge per il riconoscimento delle minoranze linguistiche rom e sinti (che vengono in parte anche dalla Croazia e di cui fanno parte 150.000 cittadini italiani, tenuti al di fuori da quello che vorremmo venisse riconosciuto ai nostri connazionali da parte di uno Stato non membro dell'Unione europea) proprio per dare la sensazione che il federalismo europeo è la risposta è la risposta e che laddove c'è la necessità di affermare i diritti di minoranze e quindi di gruppi, molto probabilmente bisogna dare *in primis* il buon esempio e poi pretendere dagli altri che si accodino.

la Croazia è per noi da tempo un partner importante, avviato con decisione sul percorso dell'ingresso nell'Unione europea. Tuttavia il nostro Paese, che ha sostenuto questo percorso in sede comunitaria, non può non subordinare ogni ulteriore passo nei confronti di Zagabria alla composizione definitiva e soddisfacente della questione degli esuli che hanno dovuto abbandonare i territori della ex Jugoslavia e a garanzie certe e a garanzie certe della tutela della minoranza italiana tuttora presente in terra croata. La mozione che abbiamo sottoscritto pone al centro dell'attenzione questi temi, che purtroppo hanno poca eco nella maggior parte dei documenti (da ultima la risoluzione del Parlamento europeo del 12 marzo scorso) e nelle notizie di stampa correlate al processo di adesione e alla diatriba sui confini con la Slovenia. I 350.000 profughi italiani residenti nei territori ceduti alla ex Jugoslavia dopo il Trattato di pace del 1947 ed i loro eredi non hanno ancora ottenuto, a distanza di più di 60 anni, giustizia per avere perso tutti i loro averi, le loro case, i loro ricordi, oltre ad avere patito la sofferenza dell'esodo dall'Istria, da Fiume, da Zara, dalla Dalmazia. Qui apro una parentesi per richiamare l'attenzione sulle responsabilità dell'Italia che, persa la guerra, ha risarcito la Repubblica Federale jugoslava con i beni degli sfollati. Il debito di guerra però è un debito nazionale e la Convenzione di Ginevra (articoli 46, 47, 53) dice che per i territori ceduti (non dal privato proprietario, ma dallo Stato) l'espropriato ha diritto a un pronto, adeguato ed effettivo rimborso, cosa che non si è mai concretizzata, tanto che come Lega Nord abbiamo presentato un disegno di legge per chiudere la questione, prevedendo la revisione degli indennizzi, finora concessi per valori irrisori (tali sono stati definiti persino dalle autorità della *ex* Jugoslavia!). Gli indennizzi sono un dovere, non un atto di generosità. L'hanno evidenziato le sezioni unite della Corte di cassazione con la sentenza n. 1549 del 18 settembre 1970, la quale afferma che in virtù della normativa internazionale (gli Accordi bilaterali italo-jugoslavi del 1949 e 1950) e di quella nazionale (legge n. 1064 del 1949) gli esuli i cui territori sono stati ceduti alla Jugoslavia avrebbero diritto al controvalore dei beni perduti secondo i principi della integralità e della proporzionalità. In attesa di riaffrontare con il Governo la questione dei risarcimenti, riteniamo sia giunto il momento di verificare con la Croazia, prima del suo ingresso nell'Unione Europea, quali siano le possibilità di restituzione di almeno una parte dei beni confiscati ai loro legittimi eredi. Mi rendo conto della portata della richiesta, ma credo che questa proposta oggi non dovrebbe più costituire un tabù, nel momento in cui la Croazia vuole essere, insieme a noi e agli altri Stati membri, parte di un'unica Comunità europea e le ruggini postbelliche dovrebbero essere ormai solo un brutto ricordo del passato.

Signora Presidente, onorevoli colleghi e colleghe, la mozione che è oggi all'attenzione dell'Aula va valutata, a mio modo di vedere, principalmente sotto due aspetti: uno riguarda il tema delle minoranze, l'altro l'entrata definitiva della Croazia nell'Unione europea. Inizierò proprio da qui per ribadire come anche la nostra parte politica sia assolutamente consapevole della necessità che questo processo venga concluso quanto prima. Si tratta di una questione che nel Friuli Venezia Giulia, e a Trieste in particolare, viene vissuta praticamente sulla pelle ogni giorno, soprattutto dopo l'entrata della Slovenia nell'area Schengen. Il confine che divide la Croazia dalla Slovenia e, indirettamente, dall'Unione europea sta diventando sempre più una ferita, una ferita profonda nel tessuto sociale, che ostacola i rapporti quotidiani, che interferisce negativamente sui bisogni delle persone ed è una zavorra per l'economia e in senso più lato per lo sviluppo globale dell'area nord-adriatica. Basti pensare alle migliaia di cittadini croati che ogni giorno varcano con non pochi disagi il confine per venire a lavorare in Italia. Mi sia consentito ricordare a questo proposito il significativo appello inviato ai Primi Ministri di Slovenia e Croazia nell'ambito di un incontro di donne svoltosi in occasione dell'8 marzo di quest'anno a Buje.

unite nel chiedere che venga definitivamente risolta la vertenza del confine sloveno-croato. Solamente all'interno dell'Unione europea sarà possibile creare in quest'area, lacerata da divisioni e dolori nel secolo scorso, un clima di civile convivenza ed integrazione. Vorrei fare presente che, solamente in questi quindici giorni di chiusura dei confini con la Slovenia a causa del G8, ci siamo potuti rendere conto nel Friuli Venezia Giulia del vero significato della caduta dei confini, del profondo valore di tale conquista per la popolazione locale. Il superamento di tutti i confini anche attraverso l'adesione della Croazia all'Unione europea darà finalmente l'ossigeno necessario per fare crescere significativamente quest'area e i rapporti tra i Paesi contermini. E allora è doveroso che anche l'Italia si impegni per dare a questo Paese il supporto necessario affinché riesca ad ottemperare a tutti gli *acquis* comunitari e a portare a compimento il processo di adeguamento agli standard europei nei diversi settori. Le recenti elezioni amministrative, svolte in un clima sereno, sono un segno tangibile che si sta procedendo sulla giusta strada. Sono convinta, inoltre, che la nuova Presidente croata Jadranka Kosor proseguirà con lo stesso impegno del suo predecessore Ivo Sanader. Ha già annunciato, infatti, di voler quanto prima concludere il negoziato con la Slovenia per la definizione del confine. Il tema della minoranza italiana in Croazia rientra nell'ambito più ampio della tutela e della valorizzazione delle minoranze linguistiche, tema di cui mi sono spesso occupata in quest'anno di legislatura. Sono pienamente d'accordo sulle richieste contenute nella mozione, ma vorrei ricordare che la Croazia, dal punto di vista legislativo, rispetta in modo corretto gli indirizzi della Carta europea delle minoranze; basti pensare ai seggi garantiti alla comunità italiana nei diversi livelli di rappresentanza, alla diffusione della toponomastica bilingue, aiuti finanziari statali per le attività culturali ed editoriali, come anche alle norme specifiche per il sistema scolastico in lingua italiana. È vero, ci sono ancora incongruenze e difficoltà in alcuni comuni che vanno superate, ma c'è soprattutto l'esigenza di mantenere vivo l'attaccamento alla propria lingua e cultura nelle nuove generazioni. In questo contesto il ruolo dell'Italia dovrebbe emergere maggiormente in chiave positiva e non con segnali poco incoraggianti**,** come il taglio operato

la presenza e il ruolo delle minoranze che vivono in quell'area plurietnica, e cioè la minoranza italiana in Slovenia e Croazia e la minoranza slovena in Italia. Dobbiamo adoperarci perché quel territorio diventi all'interno dell'Unione europea un laboratorio della convivenza e dell'integrazione, un esempio anche per quelle parti dell'Europa, dove la questione etnica è ancora è ancora motivo di scontro. Le minoranze stesse hanno dimostrato che questo percorso è possibile e ciò deriva soprattutto dall'esperienza di tanti progetti transfrontalieri positivi che insieme hanno attuato negli ultimi anni.

e la prospettiva di un ingresso in tempi rapidi nell'Unione europea, ingresso che l'Italia sostiene con convinzione, contribuiscono alla crescita di questo dialogo. Nell'ambito di questo negoziato, l'Italia sostiene pienamente i diritti delle minoranze (fra i quali quelli della comunità nazionale italiana), della Croazia all'Unione europea. L'Unione europea stabilisce che la piena garanzia dei diritti delle minoranze è un requisito essenziale per entrare nell'Unione e l'Italia svolge una puntuale azione di monitoraggio delle attività di verifica condotte a Bruxelles a tutela della comunità italiana residente nell'Istria croata

da parte del Governo croato che, a giudizio delle istituzioni comunitarie, garantisce livelli di trattamento che sono conformi all'*acquis* comunitario. Il sostegno dell'Italia al cammino d'integrazione europea di Zagabria rimane distinto dalla forte esigenza di affrontare le questioni bilaterali che sono ancora aperte in un'ottica europea condivisa. Il Governo italiano segue con attenzione le problematiche e le attese sia della minoranza italiana in Croazia e Slovenia, sia degli esuli della ex Jugoslavia. riguardo merita ricordare che si è riunito nuovamente il tavolo Governo-esuli (con due sedute, una il 5 febbraio e una l'11 giugno scorso a Palazzo Chigi, sotto la presidenza del sottosegretario Letta), che sta affrontando tutte le questioni di rilievo riguardanti gli esuli.

della restituzione dei beni appartenenti a cittadini italiani a suo tempo nazionalizzati dalla ex Repubblica Socialista Federativa di Jugoslavia. In questo spirito il Governo italiano continuerà nell'ambito del tavolo Governo-esuli e nel dialogo bilaterale con Zagabria ad adoperarsi a fondo per il superamento delle questioni bilaterali ancora aperte, in particolare quelle riguardanti i beni abbandonati. Con riferimento alla minoranza italiana che vive nei territori di tradizionale insediamento, in particolare in Istria e nel Quarnero, oltre che in Dalmazia, come è noto, attualmente essa è stimata in circa 30.000 persone. Essa si riconosce nell'Unione Italiana, che dispone di un seggio al Parlamento croato, ricoperto dall'onorevole Furio Radin, che riveste, già dalle scorse legislature, anche il ruolo di presidente della Commissione parlamentare per i diritti umani e delle minoranze. La minoranza italiana possiede una casa editrice (EDIT), una compagnia teatrale a Fiume, un centro di ricerche storiche a Rovigno, 46 comunità locali, 21 istituti scolastici e 3 dipartimenti di pedagogia. Nella regione istriana vige il bilinguismo amministrativo. Numerose municipalità istriane hanno adottato nei propri statuti comunali il bilinguismo integrale (18 complessivamente, tra cui Pola, Rovigno, Buie, Umago, Cittanova, Dignano, Parenzo), Parenzo), anche se tra grandi contrasti. Ad esempio, la toponomastica bilingue vige all'interno dei comuni, ma non nella segnaletica delle strade statali. I territori di insediamento storico della comunità italiana sono oggetto di una attenta strategia di impegno della Farnesina. Proprio per rafforzare la presenza istituzionale italiana in quei territori, oltre all'azione del consolato generale a Fiume e del consolato a Spalato, sono stati aperti recentemente due vice consolati onorari (a Pola, principale città istriana, istriana, e a Buie, centro dell'ex Zona B) e un consolato onorario a Ragusa. Per il triennio 2007-2009 il sostegno a favore della minoranza italiana in Slovenia e Croazia ha visto un impegno finanziario che nei due anni precedenti è ammontato a 4.650.000 euro annui e che per il è stato ridotto a 3.087.000 euro per i tagli nel bilancio statale. Ad esso si aggiunge l'ulteriore impegno finanziario a favore della minoranza (ex Accordi di Osimo), che ammonta attualmente a oltre 1.900.000 euro.

In occasione della prima riunione del Comitato di coordinamento dei ministri Italia-Croazia del 1° luglio scorso a Villa Madama, il ministro degli esteri Frattini ha sottolineato il ruolo della minoranza italiana autoctona in Croazia, come quella speculare croata in Molise, quale ponte tra due Paesi e due culture, importante anche nel quadro del cammino europeo della Croazia, e quale ulteriore opportunità nelle intense relazioni economico-commerciali bilaterali. In tale contesto, egli ha manifestato l'attesa che la piena tutela della nostra minoranza sia sempre garantita, in coerenza con l'accordo italo-croato del 1996 sulla protezione delle minoranze, e che, in particolare, l'attuazione del bilinguismo, prevista dagli accordi bilaterali,

per uno statuto delle minoranze. Ciò affinché il bilinguismo e la toponomastica siano omogeneamente rispettati ovunque e non vi siano differenze di trattamento delle varie minoranze. Naturalmente questo richiede un avanzamento della tutela. Mentre in Alto Adige e Sud Tirolo dopo la guerra

corso a Rijeka, è l'incultura italiana che offende i nostri esuli, la nostra minoranza, perché se la Croazia riconosce il bilinguismo in Istria, non si capisce perché in Italia non si conoscano la nostra storia e i nomi storici di quelle località. Concludendo, la volontà del Governo italiano è di consolidare la collaborazione con la Croazia, come è stato recentemente ribadito con la firma di un Memorandum di cooperazione economica bilaterale lo scorso 12 gennaio, che mira a rafforzare la cooperazione economica e industriale in settori chiave quali l'energia, l'ambiente, le infrastrutture, i trasporti, l'agricoltura, l'università e la ricerca scientifica. prima ricordato, il Ministro degli esteri ha, fra le altre cose, richiamato al collega croato la questione dei beni degli esuli, evidenziando l'opportunità, prima dell'entrata della Croazia in Europa, di trovare soluzioni che vadano incontro alle attese degli esuli in un genuino spirito europeo e nel contesto delle eccellenti relazioni tra i due Paesi. rimangono aperte questioni particolarmente impegnative, come il cosiddetto doppio voto per la minoranza italiana, l'estensione nei comuni bilingue dell'uso dell'italiano anche nei tribunali e nelle altre istituzioni pubbliche, l'aumento dei finanziamenti alle istituzioni della minoranza italiana (con particolare riferimento all'EDIT), la piena applicazione della legge sull'istruzione nella lingua delle minoranze, la continuazione dell'esenzione doganale e dell'IVA. In sostanza, il Governo italiano è fortemente impegnato nella tutela di questa minoranza, ma ma ancor più in questa azione comune europea perché tutte le minoranze possano trovare nell'ambito del Paese in cui si trovano a vivere amministrativamente il riconoscimento della loro diversità, della loro diversità, identità, storia e cultura, in un'ottica in cui esse vengano finalmente riconosciute, dopo l'epoca tragica dei nazionalismi, non come qualcosa da abbattere, ma come qualcosa da esaltare. La storia

ungheresi, slavi e italiani hanno convissuto. Il fascino incredibile di quelle realtà, che la guerra ha travolto, con un po' di determinazione, pazienza e senso della storia può essere ricostruito all'interno di un'Europa unita.

Mi permetta tuttavia di fare due osservazioni. La prima riguarda il fatto che stiamo affrontando una discussione particolarmente importante, impegnativa, che concerne non solo il futuro dell'Italia, ma quello dell'Europa. Ancora una volta siamo giunti alla conferma della scarsa sensibilità europeista di questo Parlamento e della sua scarsa sensibilità rispetto a questioni che non hanno a che fare solo con gli esuli

con la vittoria e l'affermarsi dei valori della democrazia e della libertà in tanti Paesi che non ne potevano godere. Anche la

esito di approvazione e magari anche con una partecipazione più folta dei colleghi. Al contrario, abbiamo ricercato la condivisione su questo atto, perché l'ingresso di un Paese nell'Unione europea e la tutela delle minoranze linguistiche sono questioni di dimensione storica, così come le sofferenze e i patimenti sulle terre di confine. Certo, io sottolineo in particolare ciò che hanno patito le minoranze di lingua italiana: sono storia e sofferenza della Nazione che solo negli ultimi anni hanno ritrovato diritto di cittadinanza nel dibattito storico culturale, in concomitanza,

che non ci sono, ma credo che anche la nostra valutazione comune sia molto importante. Pertanto, annunzio il voto favorevole del nostro Gruppo, con le motivazioni che ho voluto ribadire anche per dire com'è nata questa mozione: nata in sincerità, spero venga sinceramente sostenuta da tutti, e non ho dubbio che il sottosegretario Giovanardi se ne farà vigoroso e coerente interprete nell'azione del Governo della Repubblica.

che era presente (erano gli unici due di un partito di opposizione), Sovann Yim, mi ha scritto che anche nei suoi confronti è stato iniziato un procedimento di possibile revoca dell'immunità parlamentare per, ancora una volta, accusarlo di calunnia nei confronti del Governo per il semplice fatto di aver criticato, a mezzo stampa, l'operato del Governo di Hun Sen. Entrambi i senatori del partito di Sam Rainsy, dell'opposizione cambogiana, sono anche iscritti al Partito radicale non violento. Non che debba esistere una sorta di *screening* preventivo di chi entra in questo Palazzo, però se si riuscisse a coinvolgere quanto più possibile i membri della Commissione esteri in occasione di visite di parlamentari stranieri, forse

decentralizzazione o federalismo fiscale quando un politico, legalmente e legittimamente eletto, per motivi esclusivamente politici viene privato della immunità parlamentare nell'esercizio delle proprie funzioni. **Sull'applicazione della Sharia

a 40 frustate per aver indossato pantaloni sotto il normale velo islamico. Si tratta dell'applicazione della Sharia anche a donne non islamiche (non che questo faccia